Ricordo che per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato,

Signor Presidente, sarò estremamente sintetico in questa relazione. Dall'inizio di questa legislatura si è sviluppato, spontaneamente, un processo di semplificazione

Noi riteniamo che questo processo di semplificazione sia anche un processo di modernizzazione del sistema politico, da salutare positivamente. Anche per questo motivo, sono oggi in discussione presso la Giunta per il Regolamento modifiche più sostanziali e più ampie del Regolamento stesso che, tra l'altro, prevedono una maggiore corrispondenza tra i partiti, così come essi si presentano in Parlamento, e la presenza dei Gruppi parlamentari, affinché lo lo strido tra presenze alle elezioni e presenze dei Gruppi parlamentari costituisca un'ipotesi eccezionale e non la norma, come avvenuto per una parte consistente della storia repubblicana. al di là di questi aspetti (che implicano una rivisitazione del sistema politico che passa anche per le norme istituzionali e per le leggi elettorali) ve ne sono invece altri, per i quali per i quali il principio di rappresentatività resta un principio essenziale.

ha fatto presente che nel Consiglio di Presidenza, soprattutto per quanto riguarda le gestione dell'Aula, i criteri di rappresentatività hanno evidentemente il sopravvento sul criterio maggioritario che si è affermato, di fatto, nella Costituzione materiale a partire dal 1994, a noi è parso giusto aver presente questa esigenza perché, per l'appunto, si tratta di uno degli ambiti nei quali il principio rappresentativo ha certamente una sua autonomia.

corrispondenti a partiti presenti alle elezioni potessero trovare una loro rappresentanza, dovesse avere una natura di tipo transitorio. È attualmente in discussione una rivisitazione più ampia del nostro Regolamento. Sono stati nominati due relatori che stanno lavorando e hanno presentato delle proposte. Ci sembrava dunque giusto che una considerazione più generale del problema avvenisse all'interno di una rivisitazione più complessiva del Regolamento; per il momento, quindi, limitarci a prevedere solo una norma una norma transitoria che garantisse il principio di rappresentatività e che d'altra parte, però, non facesse venir meno l'esigenza naturale che questo principio non giunga a modificare il rapporto tra maggioranza ed opposizione, così come si presenta in Consiglio di Presidenza. Per questo la norma transitoria prevede anche un automatismo: laddove questo rapporto viene alterato, automaticamente il Consiglio di Presidenza si integra per consentire al principio rappresentativo di non entrare in contrasto con il principio di maggioranza; non con il principio maggioritario, che è altra cosa. Vorrei aggiungere solo un ultimo aspetto, signor Presidente, che tiene conto anche di alcune critiche che sono state formulate, soprattutto dalla stampa, sulla tendenza ad incrementare In tal senso, anche se solamente in forma si è pensato di dare una indicazione a quanti avranno il compito di operare su una rivisitazione più ampia del nostro Regolamento, evidenziando una differenziazione tra quegli aspetti che ineriscono la gestione dell'Assemblea e per i quali il principio di rappresentanza di tutti i Gruppi può essere difficilmente superato e quegli aspetti che, invece, riguardano la gestione del

Questi sono gli scarni argomenti che sorreggono

non chiude la riflessione sugli altri aspetti, come lo snellimento dei nostri lavori ed anche la creazione di organismi che siano più funzionali e magari anche più ristretti nel numero delle persone e dei colleghi coinvolti.

che finisce con il fondere due proposte, presentate, rispettivamente, dai senatori Belisario, Finocchiario, e D'Alia e dai senatori Quagliariello, Gasparri e Divina. Si tratta quindi di una sintesi delle due proposte, che cerca di attribuire alla composizione del Consiglio di Presidenza una rappresentatività che in questa legislatura mancava, evitando peraltro quegli effetti negativi che il collega Quagliariello ricordava,

ai Gruppi già costituiti. Sarà poi compito di una rivisitazione complessiva del Regolamento giungere ad una diversa e puntuale modificazione dell'istituto, che potrebbe essere valutato diversamente, proprio alla luce delle proposte di modifica presentate o di eventuali altri suggerimenti che poi i relatori già nominati per la modifica del Regolamento potranno provvedere ad effettuare. Allo stato attuale si tratta davvero di coprire un vuoto, e mi sembra vi sia grande convergenza da parte di tutti i Gruppi.

partirei proprio da questa ultima valutazione della senatrice Della Monica: si tratta davvero di coprire un vuoto o di andare a riempire un pieno? Lo dico subito in premessa perché temo di fare un intervento che non sia in piena sintonia con il Gruppo al quale appartengo. Riprendendo poi le parole del senatore Quagliariello, quando ha parlato di semplificazione o di modernizzazione, mi pongo un ulteriore dubbio:

semplicemente una spartizione, un'ulteriore moltiplicazione di poltrone, di prebende e privilegi,

che, in realtà, proprio al Regolamento del Senato stiamo lavorando perché c'è necessità di modernizzazione e di semplificazione. Se il buon giorno si vede dal mattino, auguriamoci che davvero vi sia questo processo per il prossimo il prossimo Regolamento del Senato e che invece non si vada a complicare moltiplicando ulteriormente figure e posti nuovi semplicemente per l'organizzazione e la spartizione dei posti tra i Gruppi invece che per l'organizzazione del Senato. Quindi, l'urgenza davvero non c'era visto che è proprio al Regolamento che si mette mano. Mi chiedo anche, visto che non ne è stato fatto cenno, se i senatori

porterà obbligatoriamente ad un aggravio di spese per il Senato e non mi sembra che nelle relazioni - né in quelle a voce, né in quelle scritte - vi sia alcun accenno a maggiori Lo dico visto che abbiamo da poco votato una finanziaria che interessa i cittadini che vivono fuori da questo palazzo e che hanno a che fare con i conti

si aumentano i posti, si incrementano le uscite, ma non ci si pone il problema di come coprire le spese aumentate, perché questo tema non è stato assolutamente

perché questo mi sembra davvero un po' troppo. Diciamo chiaramente che abbiamo la necessità di dare un posto in più all'Italia dei Valori perché lo scherzetto del segreto dell'urna e dell'elezione della senatrice Thaler ha prodotto questo piccolo inconveniente;

attività di studio.

Cosa è accaduto in questa legislatura? È accaduto di tutto: l'Italia dei Valori doveva costituire un Gruppo unico, poi ha deciso arbitrariamente di creare un Gruppo a parte. C'è stata probabilmente una scorrettezza all'interno dei Gruppi dell'opposizione al momento del voto da cui, da accordi, sarebbe dovuto uscire un rappresentante dell'Italia dei Valori. Ciò però alla fine non è avvenuto.

perché, a questo punto, non basta creare transitoriamente i presupposti perché anche l'Italia dei Valori sia rappresentata nel Consiglio di Presidenza:

che è stata chiosata dal primo oratore come sostenuta da scarni argomenti. Purtroppo non si è trattato di scarni argomenti, ma di affermazioni gravissime che hanno anteposto una supposta esistenza di Costituzione materiale alla certezza del diritto e alla certezza dello Stato di diritto.

Siccome quando è stata letta la relazione l'Aula non era necessariamente piena, mi prendo due minuti di tempo per leggere la relazione che è stata preparata come presentazione di questo documento, che fonde almeno tre proposte presentate nel mese di settembre e all'inizio del mese di ottobre. «L'articolo 5, nella parte in cui disciplina la composizione del Consiglio di Presidenza, é la disposizione del Regolamento del Senato che ha subito il maggior numero di interventi. Infatti, successivamente alla sua entrata in vigore nel 1971, esso è stato modificato nel 1988, nel 1993, nel 1999, nel 2001 e nel 2007». nata secondo il senatore Quagliariello nel 1994, in parte ha già visto tre modifiche di questa parte del nostro Regolamento. «Questo susseguirsi di modifiche è indice della difficoltà di trovare uno stabile punto di equilibrio tra l'esigenza di rappresentatività del Consiglio di Presidenza e la necessità di evitarne composizioni troppo ampie». per rappresentare tutto ciò che in questo Parlamento di nominati è presente. «Nella XIV legislatura, con effetto a partire dalla legislatura successiva, si è affermato il superamento del principio della rappresentanza necessaria di tutti i Gruppi parlamentari in seno al Consiglio di Presidenza».

l'assetto che si è venuto in tal modo a determinare non può ancora considerarsi del tutto soddisfacente,» - non sia mai! Siamo 322! - «in quanto del Consiglio di Presidenza non fa parte oggi un Gruppo parlamentare di significativa consistenza, espressione di una forza politica di rilievo nazionale. La presente proposta di modifica regolamentare è intesa ad ovviare a questo contingente stato di cose, salvaguardando comunque - ed in modo automatico - il preesistente rapporto tra maggioranza e opposizione». Anche in questo caso: «Tutto ciò, con una disposizione dichiarata espressamente transitoria, e quindi destinata a valere solo per la legislatura in corso». Inoltre, la disposizione medesima non varrà per i Gruppi che dovessero ipoteticamente formarsi nel prosieguo della legislatura. Anche qui: non sia mai, visto e considerato che già si sentono scricchiolare compattezze tanto nell'opposizione che nella maggioranza. Gli scarni argomenti a sostegno di questa modifica regolamentare possono essere riassunti con qualcosa che

tratta di una «modificazione tenia»: la tenia partitocratica frutto della consociazione di tutti i Gruppi e - dispiace dirlo - fatta in particolare per fare un piacere al Gruppo che ha convocato in piazza, il 5 dicembre, una manifestazione contro il Presidente del Consiglio, cari amici del Popolo della Libertà.

mano. Vedremo nel segreto dell'urna cosa avverrà. Già che ci siamo, do un consiglio per chi sta alacremente lavorando alla riforma del Regolamento: si voti per scrutinio palese, urlando il nome. E se non dovesse essere pronunciato il nome della persona desiderata, uno «scappellotto» dalla Presidenza, si torna a casa e si riprova. Perché state facendo proprio questo: un ulteriore strame della certezza del diritto nel nostro Paese. Non si tratta certo di andare a nominare il Ministro degli esteri dell'Unione europea, ancora una volta frutto della consociazione partitocratica tra PD e PdL, ma soltanto un Segretario d'Aula. Ma questa non è che l'appendice di uno stato di cose. Sarà difficile, quando si parlerà di questioni interne, andare ad individuare, grazie alla nomina, che a questo punto gli auguriamo perché sennò saremmo chiamati a votare perpetuamente il prossimo Segretario d'Aula, un rappresentante del Gruppo Italia dei Valori;

*(PdL)*. Signor Presidente, sono profondamente contrario a questa proposta di modifica del Regolamento

se fosse stato scritto, essendo una norma transitoria, che limitatamente alla XVI legislatura il Gruppo Italia dei Valori deve avere un senatore Segretario, sarei stato d'accordo; avrei votato volentieri a favore, perché di fronte ad una chiarezza espositiva mi sarei sentito appagato nella coscienza. ci si propone una prima votazione che effettivamente, come qui ho sentito dire più volte, è offensiva dell'intelligenza dei più. Ora, quando si svolgono le elezioni a scrutinio segreto, la volontà di senatori si esprime e non mi pare che si possa pensare, come ha detto peraltro la senatrice Poretti, che si sia trattato di uno scherzetto. Non è L'Assemblea dei senatori e delle senatrici decise a suo tempo un nome diverso da quello auspicato da una parte. C'è di più.

punto. Non si può dimenticare certe manifestazioni un po' estemporanee di un rappresentante di quel Gruppo che un giorno, approfittando della distrazione dei più, si è seduto abbarbicandosi su un posto riservato ai senatori Segretari dicendo che da lì non si sarebbe mosso se questo loro problema non fosse stato risolto. Ora, sotto pressioni di questo genere di solito un'assemblea nobile come questa

da parte di un Gruppo, Italia dei Valori, il cui massimo rappresentante, l'onorevole Di Pietro, si è sempre appellato al rispetto delle norme e

da parte mia. C'è una ragione in più, che è squisitamente politica: non capisco perché dovrei fare un favore al Gruppo Italia dei Valori, i cui colleghi senatori sono tutte persone rispettabilissime,

che tra l'altro, per caso, è anche Presidente del Consiglio (ma questo non c'entra), ha detto tutto quello che ha potuto dal suo veleno distillare. Allora, "cialtrone" è, e io a un cialtrone un favore non faccio.

Signor Presidente, ho ascoltato con interesse le osservazioni giunte innanzitutto dalla senatrice Poretti e dal senatore Perduca, nonché le note pervenute dal mio collega di Gruppo, senatore Longo. Senatore Perduca, non ho alcuna difficoltà ad ammettere di avere una concezione delle istituzioni differente dalla sua.

di situazioni concrete. Esse sono animate da persone in carne ed ossa e rispondono anche alle mutevoli condizioni della storia. Se lei avesse presente come si sono sviluppate le istituzioni nel mondo anglosassone, saprebbe che lì i manuali di storia delle istituzioni o di costituzionale comprendono anche discorsi parlamentari o semplici documenti, che nella materialità della situazione storica hanno comportato svolte che a volte i documenti scritti non sono in grado di determinare.

dare spazio ai risentimenti sui principi. In questo caso, è in discussione un principio che si è verificato in una situazione data: è venuto meno un principio di rappresentatività all'interno del Consiglio di Presidenza.

parlamentare, soprattutto come la concepisce lei, senatore Perduca, questo principio è sovrano. È per questo che, anche se la cosa riguarda il Gruppo più distante da noi

contro l'utilizzabilità di intercettazioni di nostri avversari, pur sapendo che un diverso comportamento avrebbe potuto procurarci un vantaggio politico. Siamo fatti di un'altra pasta: sappiamo cosa sono le istituzioni e le rispettiamo anche quando questo può non convenirci da un punto di vista politico.

credo infatti che tutto possiamo fare, tranne non chiarire esattamente qual è la questione di cui ci stiamo occupando, partendo dal presupposto che il mio Gruppo parlamentare, se avesse

Non lo facciamo solo per un atto di cortesia o correttezza nei rapporti parlamentari, ma perché siamo assolutamente convinti del fatto che questa norma serva a correggere - anche se certamente non nel modo migliore

I Gruppi più grandi, invocando un principio maggioritario che non c'è né nello spirito né nella lettera della norma (né costituzionale né regolamentare), hanno giocato all'asso piglia tutto, come si suol dire: avendo

così come prevede il Regolamento, e cioè l'Italia dei Valori ed il nostro, per evitare di alterare un equilibrio che non vi è mai stato sul piano del rapporto maggioranza-opposizione nel Consiglio di Presidenza, si è preferito eleggere nell'ambito di uno dei due Segretari il rappresentante del Gruppo Misto, perché riequilibrava sul piano dei numeri la presenza parlamentare di maggioranza e di opposizione all'interno del Consiglio di Presidenza. Questo non è nemmeno lo spirito della norma che regola l'elezione suppletiva, ma è quello che garantisce - e deve garantire - che, poiché il Senato e l'Assemblea e l'Assemblea sono la casa di tutti i parlamentari e di tutti i Gruppi parlamentari, nell'organo che li gestisce e ne dirige l'attività debbano essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari,

Questo è il dato, colleghi: possiamo discutere di tutto, ma sul piano delle regole e dell'imparzialità dell'organo che si va a rappresentare,

a non garantire nella quota dei quattro Segretari la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari: questo è il risultato. Per queste ragioni chiedo ai colleghi dell'Italia dei Valori di non accedere alla provocazione e alla tesi del ritiro della proposta e di votare, invece, per sanare questo vizio, perché quando tratta di rappresentare Gruppi parlamentari che esprimono gli elettori, gli elettori meritano sempre rispetto: anche quando essi non appartengono agli schieramenti di maggioranza o di opposizione

Vorrei ricordare che ci sono forze politiche, alle quali va tutto il rispetto - non voglio far polemica, ma bisogna parlare - che hanno evidentemente in quest'Aula e nel Consiglio di Presidenza posti di responsabilità

non un favore, ma di riequilibrare, per il diritto di rappresentanza prima più volte ricordato, la presenza all'interno del Consiglio di Presidenza, per ristabilire un rapporto di dignità paritaria tra forze politiche che hanno con orgoglio e con passione partecipato alla campagna elettorale e che si stanno distinguendo, pur nelle diversità, collega Longo, per il rispetto

le opinioni di tutti, francamente vogliamo ricordare che la presenza di una forza politica non può essere mortificata, né può essere considerata soltanto alla stregua di una di una contrattualizzazione d'Aula. Per questo ringraziamo i colleghi che hanno sostenuto la nostra richiesta, la Giunta per il Regolamento che l'ha votata, i colleghi Capigruppo, e chiediamo

mi sembra che il punto chiave di questa discussione non sia che noi stiamo creando una norma *ad hoc*, estranea allo spirito del Regolamento: il Regolamento concepisce questo organo come rappresentativo dei Gruppi parlamentari presenti in Senato. L'applicazione concreta del meccanismo del voto limitato ha violato nei fatti questo principio, perché un Gruppo (non un Gruppo qualsiasi, ma un Gruppo che corrisponde ad un preciso partito politico che ha ottenuto il voto degli elettori con quel simbolo e con quel nome) è rimasto fuori da un organo che deve essere rappresentativo. Questa è una norma che restaura

Signor Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore di questa modifica del Regolamento per le motivazioni che sono state illustrate dal senatore Quagliariello nella sua relazione. Personalmente, credo sia opportuno che tutti i Gruppi presenti in quest'Aula abbiano una loro rappresentanza in seno al Consiglio di Presidenza. Come sappiamo, ciò non è potuto avvenire perché in occasione della prima elezione, della costituzione

per quanto attento alle istituzioni e fermo sostenitore di questo Governo che pare essere osteggiato esclusivamente dall'Italia dei Valori, comunque manifesta un certo - come direbbe lui, esperto dei sistemi costituzionali anglosassoni e quindi concede (contro il Regolamento e modificandolo con una deroga che vale soltanto per i prossimi mesi) l'elezione di rappresentanti dell'unica opposizione parlamentare a questo Governo di Silvio Berlusconi. C'è un altro problema però. Sicuramente le concezioni delle istituzioni del senatore Quagliariello e le mie sono radicalmente diverse, mi verrebbe da dire. Gli suggerisco però di ricontrollare, la prossima volta che cita dei sistemi costituzionali anglosassoni, la differenza di possibilità di incidere dell'elettore attivo nei confronti del gioco e delle dinamiche politiche. In questo Paese, grazie anche a un altro obbrobrio, frutto in particolare di un autorevole esponente del Gruppo della Lega con la legge elettorale adottata nel dicembre del 2005 tutto ciò non è più possibile. Quindi, credo che la predica - diciamo professorale - relativamente alla qualità di alcuni sistemi (che non sono il nostro e verso i quali quello italiano non pare tendere in nessun aspetto del nostro vivere politico) politico) sia da confinare alle Aule parlamentari, con la speranza che qualcuno la apprezzi, la apprenda e poi la pratichi e non invece la violi dal giorno in cui gli viene chiesto di divenire legislatore. Ma in Italia i sistemi costituzionali anglosassoni sono argomento di dibattito e - ahimè - non di pratica quotidiana: la pratica quotidiana è la tenia partitocratica dell'Italia dei favori.

c'è una violazione del principio di democrazia e il mancato rispetto delle elezioni. «I Segretari... tengono nota dei senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni...» (per lo più elettroniche).

Di questo avremmo dovuto parlare e questo avremmo dovuto scrivere nel documento che ci apprestiamo a votare. Non è andata così: avete voluto presentare un'altra roba.

MARITATI *(PD)*. Ritengo che saremo più di uno a votare contro. Io voterò in dissenso dal mio Gruppo, ma poiché ci sono posizioni

il collega Quagliariello. Non posso assolutamente essere considerato in questa posizione, perché i colleghi e gli amici dell'Italia dei Valori mi sono molto vicini; condivido spesso le loro posizioni, non sempre, ma - ripeto - spesso. Quindi, non sto qui a maramaldeggiare; ma non posso accettare assolutamente il voto positivo perché esso è pericoloso. Io non ho la velleità di convincere il mio Gruppo, e neppure uno di voi: però vi invito a riflettere.

ammessa la possibilità di violare la legge sulla base di un fine buono, perché se oggi passa questo principio (per ragioni per cui peraltro non vale la pena, perché è stato giustamente detto che stiamo parlando di un Segretario), noi legittimeremo inevitabilmente la regola che, quando il fine da raggiungere è buono, si può violare la legge. La legge non si può mai violare! Questo è il principio su cui vi invito a riflettere!

Presidente, sarò telegrafico. Io non ho alcun motivo di risentimento nei confronti dei colleghi dell'Italia dei Valori. Non condivido la loro azione politica, ma questo non ha nulla a che fare con l'elezione di un Segretario d'Aula. Io voterò in dissenso dal mio Gruppo, perché sono fermamente convinto che, in un quadro di ridefinizione dell'assetto politico del nostro Paese nel senso di una tendenziale affermazione dei principi maggioritari, si debba compiere uno sforzo che alleggerisca il nostro Paese di organi che, se potevano essere assolutamente condivisi all'interno di un assetto tendenzialmente proporzionalistico, non lo sono più nell'attuale configurazione politica del nostro Paese. Ho presentato disegni di legge che prevedono che prevedono la riduzione drastica di parlamentari - senatori e deputati - di assessori, di consiglieri comunali e di componenti di sotto governo; certamente non posso operare in controtendenza relativamente a un tema come questo. Per quanto riguarda poi gli aspetti più complessivi,

fini tendenzialmente positivi. Io non credo che questo paradigma possa essere utilizzato in un caso di questo genere, né in un altro caso. La legge non può essere violata ma può essere certamente

All'interno di questo organismo, devono essere rappresentate tutte le forze politiche affinché esso, in qualche modo, operi nel pieno pieno rispetto dei Regolamenti. Io avrei allora un suggerimento da dare, se mi è permesso farlo. Questo organismo, come si diceva, è stato eletto democraticamente. Allora, senza alchimie, basterebbe che coloro i quali hanno, in qualche misura, recuperato una presenza in più la cedessero,

affinché l'organo fosse messo in condizioni di funzionare, scioglierlo e ripristinarlo con successive votazioni democratiche: basterebbe fare questo. Non c'è bisogno, quindi, di integrare l'organo con due presenze aggiuntive. Se i precedenti fanno giurisprudenza, cerchiamo di utilizzarli. Altrimenti gli organismi diventano pletorici. Mi sono spiegato? Basterebbe chiedere che chi ne ha avuto uno in più lo ceda. Mi sembra che le dimissioni siano un esercizio praticabile. Oppure

altre volte, soprattutto in sede di Consiglio di Presidenza, appoggeremo questa richiesta dell'Italia - prima il collega D'Alia ha detto "dei favori" - in questo caso dei Valori. È giusto, però, ripercorrere un po' ciò che è successo, perché questa è una storia lunga.

Voglio anche dire che l'Italia dei Valori avrebbe dovuto ottenere questo posto, se non che una faida interna all'interno dell'opposizione ha fatto sì che il Partito Democratico gli abbia "trombato" il candidato per eleggerne un altro, sempre

Gotti, Lannutti e Perduca, che tanto spesso intervengono in Aula in modo evidentemente demagogico sui costi della politica: basta! Statevene zitti una volta per tutte, perché il posto che oggi otterrete rappresenta un costo per la politica ed anche per il Senato. Dunque, coerentemente, facciamo quello che ci avete chiesto. Però, risparmiateci le vostre dichiarazioni demagogiche sui costi della politica, perché oggi voi fate esattamente il contrario di quello che in Aula da anni state dicendo.

Presidente, prendo la parola perché vorrei che fosse dissipato qualche equivoco, se non altro in ordine alla posizione del mio Gruppo che, come sapete, ha in sé anche i rappresentanti del Partito radicale. Su questo punto, nonostante l'argomento sia stato affrontato più volte anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, quindi alla presenza dell'intero Consiglio di Presidenza del Senato, mai un rilievo è venuto in ordine a quella questione posta come squisitamente politica, che è di semplicissima comprensione da parte di tutti: esiste cioè un Gruppo parlamentare con 13 senatori che non ha la possibilità o l'occasione di partecipare al Consiglio di Presidenza e, dunque, di concorrere all'organizzazione ed alle scelte politiche ed istituzionali che caratterizzano le funzioni del Consiglio di Presidenza. Una questione semplice, direi - se mi lasciate usare quest'espressione - che si inscrive tutta

significativa nel panorama politico. Quindi, francamente, non capisco cosa ci sia di così grave ed irrituale nel ritenere che nella conduzione di una legislatura - lasciatemelo dire - particolarmente significativa ed anche difficile, un Gruppo parlamentare di 13 senatori, cui corrisponde un partito con una presenza molto significativa sulla scena politica italiana, abbia una rappresentanza nel Consiglio di Presidenza. Dov'è lo scandalo? Francamente non lo capisco. Avvertivo - certamente non nel modo e nelle forme con cui lo possono avvertire il Presidente e i componenti del Gruppo

in Giunta per il Regolamento e come Presidente del Gruppo mi sono assunta la responsabilità di una proposta che ha visto coinvolti i Presidenti di tutti i Gruppi rappresentati (una proposta peraltro gestita con estrema prudenza e cautela dal presidente Schifani), per cui arriviamo oggi con questa modifica, dopo un anno e molti mesi di legislatura, a completare la rappresentanza politica piena del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. Il mio Gruppo voterà a favore.

senatore Quagliariello, è stato relatore di questa proposta. Poi si può discutere liberamente (lo hanno fatto i colleghi), perché siamo in un libero Parlamento, e nel nostro Gruppo chi ha voluto esprimere delle opinioni lo ha potuto fare.

che la Giunta per il Regolamento è un organismo particolare, non a caso presieduto dal massimo rappresentante di questa Assemblea, Sono tutti aspetti dei quali non possiamo non tener conto e che ci spingono a votare a favore. Se fossimo stati contrari lo avremmo detto prima; le ragioni ci sarebbero state, ma abbiamo preferito questa scelta di buonsenso, anche per una gestione più serena dei lavori della nostra Assemblea. Ecco perché voteremo sì, a voto palese*.

il rispetto del percorso che si sono date la Giunta per il Regolamento e la Conferenza dei Capigruppo e che è durato tanto tempo. È un percorso che si è concluso con una condivisione unanime, dopo varie articolate riflessioni, per le quali non vi era un'iniziale condivisione. Un percorso che ha visto impegnato un Gruppo di opposizione presente nel territorio, rappresentato politicamente (perché si è candidato alle elezioni politiche), ma non rappresentato in questo ramo del Parlamento. Non sta alla Presidenza del Senato, ovviamente, entrare nel merito delle motivazioni che lo hanno portato a non essere rappresentato, ma ciò era un dato di fatto. Vi sono state fortissime lamentele da parte di questo Gruppo, che ha lamentato l'assenza di rappresentanza. Questa Presidenza ha cercato per un certo lasso di tempo di per trovare una soluzione e contemperare questo problema - che tocca anche il contenimento dei costi - con quello della rappresentanza.

È evidente che ciò va a toccare temi di altro genere, quali l'eventuale aumento dei costi. Vorrei segnalare ai colleghi, come, grazie all'intervento dei senatori Questori ed anche alla condivisione dei nostri bilanci, questo Senato ha ha da tempo, sin dal mio predecessore, presidente Marini, iniziato un'opera di riduzione e contenimento dei costi, che ha toccato le missioni (anche quelle internazionali) i benefici e l'aspetto pensionistico, con la riforma iniziata con il presidente Marini. Abbiamo iniziato un percorso e continueremo ad essere sempre più attenti e rigorosi: posso esserne garante, nella consapevolezza di avere il conforto dell'intera Assemblea, così come ho sempre avuto il conforto dei senatori Questori che rappresentano sia la maggioranza che l'opposizione.

l'andamento della spesa del Senato, tenuto sotto controllo dai senatori Questori, va sempre nel senso della riduzione dei costi complessivi della macchina del Senato.

25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010***

insisto su un argomento che non può non stare a cuore. È da questa mattina che ci sentiamo dire che i nostri

cicli. Se una famiglia spende più di un terzo dello stipendio di un capofamiglia per i libri di testo del primo anno di liceo, forse chiederà al figlio di non frequentare il liceo. Può il Paese rinunciare a talenti e a persone che potrebbero continuare gli studi fino all'università? La maggioranza vuole qualificarsi sul fatto che l'uso della tassa non deve essere punitivo.

Spiace che il relatore, questa mattina, abbia dovuto presentare, prima ancora che illustrassimo i nostri emendamenti, un ordine del giorno che dal suo punto di vista avrebbe sintetizzato,

La sede parlamentare è la sede propria per far emergere l'unità sui temi che ci stanno davvero a cuore. Consentire la prosecuzione degli studi ai meritevoli e ai capaci, in particolare dove borse di studio non ce ne sono più, è possibile solo attraverso il meccanismo della detrazione. Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi affido di nuovo alla vostra riflessione, avendo già acquisito un parere contrario,

Ricordo allo schieramento che di solito è il paladino della parità scolastica che mancano 135 milioni di

allora perché non approvare l'emendamento 1*-bis*.0.1, visto che poi tutti gli ordini del giorno fanno la stessa fine. comunali, cattoliche, laiche, comunque riconosciute dallo Stato abbiano una funzione pubblica, soprattutto verso i più piccoli, e allora votate questo emendamento; oppure cominciate a suggerire al Ministro

che si chiama - o è stato chiamato, in maniera strumentale - «salvaprecari» e scopriamo che in realtà sana solo in piccolissima parte un danno che lo stesso Governo ha procurato a tante decine di migliaia di insegnanti. Forse dovremmo smettere, signor Presidente e caro Sottosegretario, di chiamare queste persone «precari»: in quest'anno di dibattito siamo, o meglio, siete

(la prendo un pochino alla larga, ma per fortuna abbiamo qualche minuto). Credo anche si debba cominciare ad essere riconoscenti a tante decine di migliaia di persone

finanziamenti aggiuntivi e sanare una situazione complicata: lo facciamo per la scuola pubblica e per i tanti precari, perché abbiamo a cuore il futuro del nostro Paese. Quindi riteniamo che gli investimenti nella cultura, nella formazione, nella scuola, nella ricerca e nell'università siano prioritari. E abbiamo la coerenza di farlo anche rispetto alle scuole come diceva poc'anzi il nostro Capogruppo in Commissione, senatore Rusconi. Il Governo

delle normative di legge che il precedente Governo, il Governo Prodi, aveva voluto con la finanziaria 2007. Parimenti, questo Governo e questo Ministro in tante sedi e in maniera ripetuta si dichiarano paladini delle scuole paritarie, dicendo di volerle finanziare e di riconoscere l'attività sociale che viene svolta dalle scuole comunali, sia nei grandi centri come Milano sia in quelli piccolissimi, dove spesso esse sono l'unica istituzione scolastica presente quelle comunali, a quelle cattoliche e a quelle laiche). Ebbene, almeno si abbia il coraggio di gettare il velo, di chiarirsi e di essere trasparenti - diciamo così - nei confronti dell'opinione pubblica. Noi questo velo lo gettiamo chiedendo di votare a favore di questo emendamento e di ripristinare questi fondi per le scuole paritarie, così come abbiamo chiesto di ripristinare i fondi a favore dell'istituzione scolastica pubblica.

che è l'unico strumento che consente di avere, in modo nominativo, il quadro dei ragazzi che abbandonano il percorso scolastico o che hanno comunque un numero di bocciature tale da portare alla dispersione e all'abbandono della

2, in modo assolutamente improprio si propone invece di inserire all'interno dell'anagrafe scolastica, che deve essere puramente nominativa, dati molto sensibili dal punto di vista personale, primo fra tutti la valutazione dei ragazzi,

**Il Senato non approva.**

''Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno

ma è una misura d'urgenza - l'ennesima - che cerca di rimediare a problemi che si sono presentati all'inizio dell'anno scolastico anche, e purtroppo, a causa dei grandi tagli finanziari che ha dovuto subire il settore della scuola e, in particolare, il finanziamento degli insegnanti.

devono affrontare tale mercato del lavoro più difficile e concorrenziale con una scuola che purtroppo non è all'altezza di quello che richiede il mondo stesso. Mancano fondi e purtroppo in questo settore il Governo ha dimostrato finora poca sensibilità; mancano la volontà e il sostegno politico Signor Presidente, colleghi, non per autocompiacimento ma perché penso che si possa seguire quale esempio, vorrei ricordare che, a differenza del resto del territorio nazionale, a Bolzano, a Trento e in Valle d'Aosta viviamo per fortuna una situazione completamente diversa. Abbiamo avuto i migliori risultati nelle valutazioni PISA, non solo in confronto alle altre Regioni d'Italia ma a livello europeo. La scuola, in particolare per quanto riguarda la nostra Provincia, quella di lingua tedesca, grazie ad una più ampia autonomia si è potuta piazzare ai massimi vertici della valutazione PISA, allo allo stesso livello della Finlandia che si trova al primo posto. Questo risultato riguarda la scuola dell'obbligo e le scuole secondarie,

a una qualificazione e a una professionalità di altissimo livello, che permettono di entrare nei vari settori, dall'artigianato, al turismo, al mondo industriale, disponendo di una preparazione e non solo di un titolo di studio.

le considerazioni che vorrei trarre, la prima è di prevedere, in una riforma che auspichiamo arrivi presto, un sistema più regionalizzato, cioè più vicino alle Regioni e alle Province, anche per gli insegnanti, chiedendo loro di essere residenti,

siano effettivamente scelti i migliori. Penso al sistema inglese e a una modalità di selezione con la quale il direttore didattico abbia la responsabilità e l'autonomia di valutare personalmente le qualità degli insegnanti e di scegliere la migliore soluzione per la propria scuola. luogo, occorre un sistema di valutazione continua dell'insegnamento stesso e degli insegnanti, del quale si tenga conto, e una valutazione del sistema scolastico italiano l'istituto INVALSI che riferisca i risultati delle prove non solo a una pura statistica nazionale e al raffronto alle varie Regioni e Province ma tenga conto dei risultati di queste prove anche per valutare gli stessi insegnanti.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la discussione che si è accesa negli ultimi due mesi sul decreto salva precari e che ora giunge, forse, alla conclusione merita qualche riflessione più attenta soprattutto per i non addetti ai lavori e per tutti coloro i quali pensano o sono convinti che questo provvedimento metterà a posto il subbuglio venutosi a creare nella scuola in seguito alla impropriamente detta riforma Gelmini, che altro non è che uno scriteriato taglio al personale e all'offerta formativa della scuola. Se solo oggi ci troviamo a parlare dei precari e su come salvarli è perché, evidentemente, c'è un problema, e grande; è come al solito, si è dovuti correre in fretta e furia a mettere un riparo, a tamponare un disastro che una superficiale e cinica riforma ha creato; è perché, per forza di cose, si è dovuto riconoscere che esistono della persone in grandissima difficoltà economica ed esistenziale. Sarebbe persino inutile in questo momento soffermarsi sul disagio che stanno attraversando tutti gli ordini di scuola, dalle elementari alle scuole superiori, quando si decide, esclusivamente per fare cassa, di sottrarre 8 miliardi di euro alla pubblica istruzione e di calare dall'alto una riformetta varata nel bel mezzo dell'estate. No! Qui bisogna sottolineare con forza la violenza esistenziale che una cattiva politica sta perpetrando ai danni di una categoria, quella degli insegnanti impropriamente detti precari, che prima di tutto sono persone umane con una loro dignità e un diritto al futuro. Quando si decide di dire sì oppure no, cari colleghi, è doveroso mettersi davanti agli occhi questa realtà, usare la coscienza per rendersi conto di quanto le nostre decisioni possano persino compromettere la possibilità per delle famiglie di mangiare, di fare la spesa decorosamente. Non dobbiamo raccontarci frottole per tacitare il fatto che questo Governo e questa maggioranza lascerà senza reddito nel prossimo triennio 150.000 persone, che diventano più del doppio se consideriamo le famiglie che contano su quel reddito, e che la scure quest'anno ha già lasciato a spasso 42.000 fra personale docente e ATA. Qualcuno, forse, ce l'ha fatta *in extremis* ad avere qualche supplenza; altri, la maggioranza, non hanno visto rinnovato il proprio contratto di lavoro. Da questi numeri spaventosi nasce l'urgenza del salva precari, non da altro! Ma poi ci si chiede: ma chi si sta salvando, e da cosa? Ee perché? Come ho appena detto prima, questi docenti li si chiama impropriamente precari per sminuire il problema, per rendere più asettica e chirurgica la loro eliminazione: di questo stiamo parlando. Tanto per cominciare, quando un docente entra in classe, sia esso precario o di ruolo, assume formalmente le stesse responsabilità, gli stessi obblighi, gli stessi doveri; anzi, gli obblighi sono i medesimi, i diritti un po' meno. Per chi non lo sapesse, questi docenti negli ultimi dieci anni, ma in moltissimi casi anche da molto più tempo, hanno mandato avanti le scuole, soprattutto in luoghi lontani e in sedi spesso disagiate, al prezzo di grandi sacrifici personali e familiari; sono stati presenti nelle commissioni d'esame, si sono specializzati attraverso *master* e seconde lauree, tutto a proprie spese, e potremmo continuare l'elenco. Ora cosa si fa? Siccome la coperta si dice essere corta, il più forte trova più semplice la lotta con il più debole, e così si inventa una serie di bugie per screditare queste persone e gettarle via. Vorrei dire che per questi docenti la scuola non è stata un ammortizzatore sociale: anzi, è vero il contrario, perché è stata la scuola ad utilizzare questo personale per anni e a sfruttarlo con il minimo dello stipendio, senza alcuna possibilità di ricostruzione della carriera i relativi scatti di anzianità, licenziandolo a giugno per riassumerlo a settembre, reiterando i contratti a tempo determinato e abusandone. In questo modo si diventa precari anno dopo anno, quando lo Stato sfrutta il lavoro altrui, quando lo Stato rinvia decisioni e lascia incancrenire i problemi che poi si lasciano pagare, senza pensare alle conseguenze, a persone che non si possono difendere. Per capire realmente di cosa ha bisogno la scuola bisognerebbe entrarci dentro, viverla con questi professori, farsi raccontare le loro esperienze, utilizzare la loro esperienza affinché il servizio e l'istruzione possa innalzarsi e competere a livelli europei. Non possiamo lasciare per strada questi insegnanti che, legittimamente, speravano, e continuano ad avervi diritto, ad un posto di lavoro certo e stabile. Vorrei rivolgervi una domanda: ma se a quarantacinque anni ci dicessero che, dall'oggi al domani,

Se a questo aggiungiamo tutto ciò che fa capo ad una famiglia sentiremmo il peso della sopravvivenza. La posta in gioco è questa, ed a nostro avviso è altissima. Il cosiddetto salva precari, in realtà, non salva niente e nessuno, lascia agonizzare migliaia di persone per due anni con l'elemosina di un sussidio di sopravvivenza, lasciando le porte del futuro spalancate sul baratro: questa è la verità per noi dell'Italia dei Valori. Il salva precari avrebbe potuto essere una valida soluzione tampone solo se il Governo avesse mostrato l'intenzione di tornare sui suoi passi, fermarsi un attimo e riconsiderare l'ottica dei tagli, e dare a questi insegnanti ciò che legittimamente chiedono: il loro posto di lavoro. Se ci fosse buona volontà potremmo tutti insieme fare qualcosa proprio su quest'ultimo punto: il blocco dei tagli per i prossimi due anni, in modo da restituire speranza a questa gente. Guardate, colleghi, non possiamo girare la testa dall'altra parte e far finta che questi professori e il personale ATA non esistano: esistono eccome. Vi invito a fare un giro sulla rete, a visitare i *blog* ed i vari siti dedicati a questo argomento: vi renderete conto che ci sono tante storie vive, piene di paura e rabbia, in attesa che noi politici ci accorgiamo di loro e dialoghiamo dialoghiamo con loro; altrimenti, tutti avremo fallito e disonorato il nostro mandato. In quest'Aula voglio denunciare un altro fallimento, quello dell'informazione, che ha reso la protesta dei professori precari invisibile e, dunque, inesistente. Infatti, in questo mondo fatto di apparenza e tv, ciò che non appare, di fatto, non esiste. Porto un esempio per tutti: dal 1° settembre 2009 il centro servizi amministrativi (CSA) di Catania è occupato ininterrottamente, di giorno e di notte, quindi ventiquattr'ore al giorno, da questi insegnanti e dal personale ATA; questa gente dorme lì, trascorre lì le giornate, facendo turni, organizzando manifestazioni e *sit-in*. Nessuno se ne è accorto. A Palermo ed a Messina c'è stato uno sciopero della fame: ne avete saputo niente? Qualcuno di voi è andato lì? Noi ci siamo stati, signor Presidente. O davvero serve sempre e solo l'azione eclatante e scioccante per far sì che un cittadino possa sottoporre all'opinione pubblica la sua sofferenza ed il suo disagio? Noi dell'Italia dei Valori concordiamo con il personale della scuola quando afferma che siamo in presenza del più grande licenziamento di massa dell'Italia repubblicana, che avrà conseguenze più dure e devastanti nelle Regioni del Meridione.

Nessuno di noi, tanto meno i ministri Gelmini e Tremonti hanno il diritto di entrare così pesantemente nell'esistenza della gente, condizionarla così tanto da azzerarne il futuro. Infatti, quando si nega ad un individuo la possibilità di un progetto, tutti voi in quel momento lo state uccidendo, state commettendo un vero crimine. Il Governo non può facilmente e pilatescamente lavarsene le mani addossando come scusa questo problema a chi l'ha creato. Volendoglielo concedere, il ministro Gelmini non può esimersi dal dare a questa gente, lei per prima, una risposta non ideologica: a questi insegnanti non interessa per niente essere etichettati in uno schieramento politico; non possono permetterselo, perché devono sopravvivere. Un vostro sì a questo decreto ha il potere devastante di compromettere il presente e il futuro di queste persone. La saggezza deve spingerci a ritornare sui nostri passi, poiché decisioni affrettate, in malafede o frutto di clientelismi di bassa lega ledono e negano lo Stato di diritto. In questo decreto imbroglia precari si è voluto inserire, di sponda, una modifica che riguarda direttamente la Sicilia, e precisamente il concorso regionale per dirigenti scolastici finito al Consiglio di giustizia amministrativa, oltre che sui giornali e in televisione. Ricordo brevemente la storia di questo concorso: bandito con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, era stato annullato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decisioni inappellabili, signor Presidente, pubblicate il 25 maggio 2009, nn. 477 e 478. Nonostante le sentenze, la graduatoria era stata approvata e i vincitori nominati. Ora, un emendamento proposto dalla maggioranza, da voi, vuole risolvere il contenzioso in corso relativo alle procedure concorsuali praticamente con una sanatoria, poiché l'emendamento, nei fatti, prevede che l'annullamento degli atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del decreto n. 140 del 2008 non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio. Ovviamente questo è un altro *escamotage ad personam* che viola il dettato costituzionale in quanto fa riferimento ad un concorso invalidato dal Consiglio di giustizia amministrativa; come appare banalmente ingenua la motivazione di chi vorrebbe farci credere che in questo modo si tuteli il corretto avvio dell'anno scolastico! Oggi il Governo in Aula, anziché eliminare questa indecente sanatoria, ci fa sapere che porterà un provvedimento per annullare il concorso e per sopprimere la sanatoria la sanatoria prevista alla Camera dei deputati. Noi dell'Italia dei Valori, signor Sottosegretario, avevamo offerto la disponibilità a cambiare durante l'esame in Aula questa imbarazzante situazione che certamente evidenzia profili di incostituzionalità del provvedimento. A noi tutto ciò sembra un'ulteriore violenza e beffa a danno dei precari che, legittimamente e onestamente inseriti in una graduatoria ad esaurimento, continuano a restare in fila in attesa del loro posto di lavoro. Per tutto quello che ho detto e per quanto

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il decreto sui precari annulla alcune sentenze del TAR, imponendo che i supplenti della scuola siano inseriti nelle graduatorie secondo le modalità precedentemente stabilite dal Ministero (in pratica, per il periodo 2009-2010 è il blocco dei trasferimenti), evitando così il caos. Rimane naturalmente il problema del 2011, quando ci si potrà spostare da una provincia all'altra col riconoscimento del punteggio, in certe zone spesso acquisito in maniera tutt'altro che cristallina. Per questo, in attesa della riforma del reclutamento in senso regionale ed accogliendo l'appello dei tantissimi insegnanti precari onesti che temono di vedere ridotte al lumicino le possibilità di trovare ancora spazio nel mondo della scuola, abbiamo presentato un ordine del giorno, che il Governo si è impegnato a trasformare a breve in un atto concreto, con cui chiediamo, nel caso di trasferimento di provincia, la revisione dell'attribuzione dei punteggi. Inoltre, a partire dalla prima integrazione delle suddette graduatorie ad esaurimento, i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado dovranno essere valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio che, in mancanza di tale certificazione, non potrà essere valutato. Puntiamo in questo modo a stoppare il fenomeno dei docenti che figurano aver lavorato, pur non avendo in realtà mai messo piede a scuola (notoriamente ci sono docenti che pagano per avere la certificazione di servizio) e quello dei docenti che lavorano gratis o quasi e senza contributi, pur di avere il punteggio. punteggio. Questo è solo il primo passo, perché gli insegnanti rispettosi delle regole, che dal 2011 rischiano di trovarsi sulla strada, giustamente reclamano a gran voce la completa verifica della veridicità degli esorbitanti punteggi acquisiti da certi colleghi. Il Governo si è anche impegnato a correggere l'articolo del decreto che sana la posizione dei dirigenti scolastici della Sicilia in esito al corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione del 22 novembre 2004, nel quale si sono evidenziate una serie di irregolarità. Per tutti questi motivi la Lega Nord esprimerà voto favorevole al provvedimento.

non casualmente: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».

Al di là dei titoli, il risultato è che su ogni provvedimento della scuola italiana da un anno e mezzo sovrasta la tagliola o, meglio, la clausola di salvaguardia dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, ovvero come si tagliano otto miliardi di euro sulla scuola italiana, dopo che il Ministro a più riprese in questo anno ha detto più volte che i tagli per il 2010 erano solo indicativi e che sarebbero cambiati in finanziaria. La finanziaria è già passata da quest'Aula e nessuna nuova buona notizia è arrivata. Si è affermato da parte del relatore e della maggioranza

Bastava accettare qualcuno dei nostri emendamenti, invece di blindare il provvedimento, e ne avreste aiutate 30.000. Voglio chiedere alla maggioranza e al Governo: secondo voi, questi docenti avrebbero preferito essere aiutati o essere assunti? Bastava non boicottare e non sospendere nei fatti il piano triennale della finanziaria 2007,

alla Camera, Valentina Aprea, ritenne quel provvedimento insufficiente per i precari: non era abbastanza per dare risposte efficienti alla gravità della situazione dei precari italiani.

C'è un dato, a mio parere, che è estremamente grave: avete cambiato le regole dell'assunzione di queste persone a gara in corso, a metà percorso. percorso. Con la finanziaria 2007, che prevedeva delle graduatorie a chiusura dopo tre anni, questi docenti hanno scelto di rimanere o di non rimanere nella scuola di rimanere o di non rimanere nella scuola calcolando se entro il 2010 sarebbero entrati in ruolo o meno. Hanno, quindi, deciso di rimanere nella scuola perché sarebbero stati assunti a tempo indeterminato.

che avreste accettato un ordine del giorno. Sembra che non abbiate altre risposte. Addirittura, come ha detto bene prima il collega Giambrone, rispetto a un provvedimento della magistratura amministrativa che dichiarava chiaramente nullo

pur di fronte al dato reale che il concorso era nullo, le persone e i dirigenti scolastici che erano risultati vincitori e avevano ottenuto il posto salvavano quel posto;

Avete fatto la stessa cosa con le scuole paritarie, voi che siete i difensori della libertà educativa, più di noi. In realtà non

risposto? Ci avete risposto con un ordine del giorno. Ma fidandovi dei vostri ordini del giorno le scuole paritarie aspettano ancora i 120 milioni di euro dell'anno scorso, come il Ministro mi ha puntualmente confermato venti giorni fa rispondendo ad un'interrogazione a risposta scritta.

Peccato che avete detto la stessa cosa anche rispetto alla nuova legge sull'università, ai finanziamenti alle scuole statali per il 2010 e ora lo dite anche rispetto alle scuole paritarie.

A me sembra che le famiglie e la scuola italiana aspettino risposte serie.

ha confermato che i titoli migliori su cui investire per ottenere rendimenti elevati non sono le azioni o le obbligazioni, ma i titoli di studio: diplomi, lauree e *master* rendono di più, nel lungo e nel medio termine.

contrariamente a quanto sta avvenendo in Italia, il programma del nuovo Governo tedesco prevede, nell'arco della legislatura, un incremento della spesa per l'educazione e la ricerca di ben 12 miliardi di euro.

un piano triennale di assunzione di 150.000 precari, di personale ATA, la chiusura delle graduatorie e un piano di incentivazione ed assunzione di giovani nella scuola.

Colleghi, sono presenti in tribuna alcuni studenti nell'ambito del progetto di gemellaggio tra una scuola per sordi dell'Ohio

Vorrei ricordare a me stesso, ma soprattutto ai colleghi, che in quel periodo i docenti precari rappresentavano il 50 per cento del corpo docente e dunque oltre mezzo milione di persone.

che ha creato una degenerazione, dando l'illusione a tanti laureati di poter entrare nei ruoli della scuola.

di avere comunque un ammortizzatore sociale importante, poiché circa 18.000 persone non si troveranno senza stipendio. Non solo, costoro avranno diritto al punteggio

del posto fisso e del posto sicuro. È ora di finirla, anche e soprattutto nel mondo della scuola. Signor Presidente, nessuno ricorda che in questo Paese spendiamo quanto la Finlandia per ogni studente: 5.700 euro all'anno. Ebbene, abbiamo la stessa scuola della Finlandia? Assolutamente no, perché abbiamo un terzo di insegnanti in più e problemi immani, perché il grosso della spesa serve solamente per gli stipendi dei nostri docenti. Allora, dobbiamo riparametrare tutto e rivedere le posizioni. Con il riordino che ci apprestiamo

è l'errore più grande che questo Paese ha fatto per anni, ed è ora di finirla: ebbene, anche su questo decreto, che è minimale e serve solamente ad aiutare i deboli,

per il futuro bisogna evitare la situazione in cui si trovano oggi migliaia di precari, in fila da troppi anni in graduatorie infinite e alle prese con l'accumulo di punti che consentono loro di scalare di posizione e ottenere la nomina chissà quando. Allora, ha fatto bene il Governo ad interrompere e arginare una situazione che rischia ormai di incancrenirsi e far precipitare nel baratro il governo della scuola: per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di individuare le migliori soluzioni possibili per sanare la situazione che abbiamo ereditato. Con il provvedimento che oggi esaminiamo vogliamo rendere operative le immissioni di urgenza, per risolvere la situazione transitoria dei precari che per l'anno scolastico 2009-2010, come dicevo, non si troveranno nelle condizioni di veder rinnovato il loro contratto annuale. però, questo Governo non vuole limitarsi ad una visione di breve periodo, ma intende agire in profondità, riformando il reclutamento e la formazione iniziale e dotando gli insegnanti italiani come tutti quelli europei - questo sì - della carriera

che mi auguro possano trovare in Parlamento soluzioni ampiamente condivise. Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro in maniera convinta il voto favorevole del Popolo della Libertà al provvedimento in esame.

e che sia accettabile una discussione sul tema dell'immigrazione clandestina, ma ciò che non è accettabile è teorizzare e praticare la pulizia etnica.

e l'ordinamento vigente, di scioglimento degli organi di quel Comune del bresciano, ed è motivo per aprire un procedimento penale a carico degli amministratori per istigazione all'odio razziale. per istigazione all'odio razziale.

ne siamo certi e aspettiamo fiduciosi. La seconda questione, e concludo, signor Presidente, riguarda la visita del leader libico Gheddafi in occasione del vertice della FAO. Abbiamo letto tutti sui giornali che, in ossequio al suo credo religioso, il leader Gheddafi ha organizzato due festicciole con avvenenti ragazze - selezionate, secondo un sistema di *casting*, per per età, abbigliamento, taglia, altezza e quant'altro alle quali sarebbe stato regalato anche un Corano, circostanza che non ha prodotto alcuna protesta da parte di chi ritiene che il Corano non debba essere diffuso in questo Paese. Ma ciò che a me più interessa di questa vicenda, poiché credo che la rappresentazione di questi fatti e il modo in cui il leader libico si è comportato sia offensivo

è un Paese serio e non un Paese nel quale un leader come Gheddafi può permettersi di venire ad insultare le donne, così come ha fatto in due circostanze.

A nome del Partito Democratico chiediamo al Ministro dell'interno di venire il più presto possibile a riferire in Aula in merito all'iniziativa intrapresa dal sindaco e da tutta la giunta del Comune di Coccaglio, un Comune in provincia di Brescia che ha visto crescere negli ultimi anni la popolazione immigrata. Questo è un dato oggettivo. [**Presidenza della vice

Non vorremmo che a distanza di millenni il nostro Paese, riconosciuto nel mondo come difensore e propugnatore dei diritti umani,

(che poc'anzi ha detto che i senatori Lannutti, Pardi e Li Gotti d'ora in avanti devono fare attenzione a muovere critiche al Governo e alla maggioranza), mi permetto di segnalare le insufficienze e i disservizi che hanno interessato il passaggio dall'analogico al digitale terrestre,

hanno visto nulla per l'intera giornata, ma si sono anche dovuti improvvisare tecnici per sintonizzare i canali, senza alcun esito. A pagare lo scotto maggiore di questa lodevole, seppur malgestita, innovazione sono stati gli anziani non in grado di far fronte a un cambio di tecnologia così complicata e sofisticata. Oggi, a pagina 32 del

Pochi minuti fa, ho voluto parlare con il sindaco di Coccaglio, che mi ha testualmente detto: ma come, applicare le leggi che il Parlamento approva vuol dire essere lesivi dei diritti umani? Lo chiedeva a me, in qualità di senatore che ha votato e voluto quella norma che ha ridotto a sei mesi il termine per la cancellazione anagrafica degli stranieri che non rinnovano la dichiarazione di dimora abituale dopo che è scaduto il loro permesso di soggiorno. Si tratta di una procedura di cancellazione anagrafica prevista da una norma di legge

È una procedura codificata da una legge, e non c'è nessun intento persecutorio. Il problema è che ci sono sindaci che applicano le leggi e sindaci che non vogliono farlo perché la loro ideologia le loro convinzioni culturali li portano a non applicare delle leggi votate democraticamente dal Parlamento. Ripeto: non c'è nessun intento persecutorio. La denominazione «White Christmas» è una denominazione giornalistica che non trova riferimento in nessun atto di quella amministrazione. Stiamo parlando di un'amministrazione che doverosamente ha fatto quello che io, per esempio, come sindaco, e tanti altri sindaci abbiamo già fatto nel corso degli anni passati. La differenza è che prima dovevamo attendere un anno - questo era il termine fissato nel 1989 - mentre adesso l'abbiamo portato a sei mesi, e cerchiamo di accelerare i tempi. L'unica pulizia che si sta facendo è una pulizia anagrafica anagrafica), non etnica, non di razza. Stiamo facendo ciò che un amministratore serio deve fare. Concludo facendo un'affermazione, perché ho sentito parlare prima del reato di istigazione all'odio razziale. Il senatore D'Alia diceva di sperare che questo sindaco venga

di divieto di parlare per tre anni è un fatto che in una democrazia normale non dovrebbe mai accadere! Possiamo scontrarci e avere opinioni diverse, ma mai mettere la sordina ad un uomo per tre anni!

cui lui si richiamava, richiede anche il rispetto del codice, che prevede che l'istigazione all'odio razziale sia

signora Presidente, io ho preso la parola per un'altra questione. Oggi un autorevole quotidiano, il "Corriere della Sera", ha dedicato ben due pagine centrali allo scandalo che interessa la mia Regione, la Lombardia, e che riguarda le aziende del ragionier Giuseppe Grossi, attualmente detenuto a San Vittore per reati reati fiscali, appropriazione indebita e riciclaggio, collegati alle bonifiche di alcune aree, la più famosa delle quali è quella di Santa Giulia a Milano.

dal dottor Resca, attualmente direttore generale del Ministero dei beni culturali, chiamato dal ministro Bondi a svolgere questa funzione,

il dottor Resca ha provveduto a dismettere uno zuccherificio e, con i proventi di questa dismissione, a realizzare un'altra attività industriale per la quale la società

Come direttore generale di un Ministero e, quindi, come rappresentante del Governo o come portatore di un interesse specifico, che voglio sperare legittimo? **Sulla

ha legato le lenzuola e si è impiccato all'inferriata. Era stato arrestato per un tentativo di furto con un cacciavite in una stazione della Lunigiana, dove lavorava come operaio. Rilevo soltanto che, se fosse stato italiano, il diciassettenne avrebbe avuto sicuramente, per quel tipo di reato, gli arresti domiciliari. Aveva la sventura di essere marocchino e per lo stesso reato è stato in carcere alcuni mesi, fino a che la sua mente non ha più retto la situazione. Chissà cosa avrebbe potuto fare quel diciassettenne se non avesse deciso di ammazzarsi!

al giudice Meucci che è stato uno degli inventori del diritto minorile. Egli è ricordato dappertutto, non solo in Toscana, come il codificatore di un atteggiamento nei confronti dei minori che si sono si sono caratterizzati per reati, sulla base di un approccio severo ma umano, profondamente inteso alla prassi del recupero. Evidentemente il nome di Meucci sta impigliato sull'architrave del carcere, ma non è stato sufficiente a convincere il giovane diciassettenne a vedere in quel carcere l'umanità che pure il suo nome promette.

Spero, però, che quando verrà restituito il favore - perché ormai costui è un partner strategico - anche magari dal prossimo Ministro dell'Unione europea non venga consegnata la Bibbia al posto del Corano. **Sui